L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Esistono - è vero, è stato detto - delle realtà oggettive e sociali da combattere come il lavoro nero, settore in cui ci sono più infortuni perché c'è meno prevenzione. Lo stesso vale per la frammentazione del lavoro, le squadre, i subappalti e il problema delle piccole imprese.

Gli incidenti avvengono sempre nell'ultima spedizione e nell'ultimo momento della giornata, quando l'attenzione declina. La formazione va fatta sull'aspetto del rischio e sulla consapevolezza del rischio che i lavoratori devono avere perché certi comportamenti vengano mantenuti costanti nell'arco della giornata: quando uno è stanco e non ce la fa deve smettere di lavorare.

il decreto legislativo n. 106 del 2009 ha sostanzialmente abrogato. Come ho detto questa mattina e come ripeto oggi nella dichiarazione di voto,

ad ottenere un po' di ordine, e magari anche che alcuni dialoghi necessari e indispensabili si svolgano fuori dall'emiciclo.

per l'Italia dei Valori è importante che per combattere il fenomeno degli infortuni sul lavoro ci sia un doppio binario: un regime sanzionatorio, importante per quei datori di lavoro che non investono nella sicurezza nelle loro aziende e che violano la normativa antinfortunistica,

il regime sanzionatorio precedente, rendendolo di fatto inefficace. Questa mattina ho sentito dire dal Sottosegretario, con con una frase un po' nebulosa, e in politichese, per così dire, che si avvierà un percorso per capire qual è il punto di mediazione fra il precedente regime sanzionatorio e quello attualmente in vigore. Prendiamo atto dal Governo che si avvierà questo percorso e sicuramente la Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro darà il proprio contributo, ma ad oggi oggi non ci sentiamo di approvare una risoluzione in quest'Aula dove non si preveda l'impegno del Governo a ripristinare il sistema sanzionatorio previgente. Dopodiché, vedremo quale potrà essere eventualmente il punto di mediazione, ma ad oggi questa è la nostra posizione. Dico questo anche perché è evidente che quando parliamo di

quindi che il momento sanzionatorio, anche per creare una cultura della legalità e del rispetto della normativa antinfortunistica, sia importante.

Presidente, colleghi senatori, la difficoltà che il gruppo di lavoro da me coordinato sta incontrando è la dimostrazione della necessità, da più parti sollevata nel corso dell'attività della Commissione e richiamata dal presidente Tofani, di un maggior coordinamento tra i vari enti competenti in tema di prevenzione e vigilanza. Lo stesso ministro Sacconi, nelle audizioni del 7 e del 14 ottobre dello scorso anno, ne ha sottolineato la necessità, unitamente a quella sulla raccolta unificata dei dati e l'avvio di campagne di formazione e informazione. A dimostrazione di quanto appena detto, per quanto riguarda il gruppo di lavoro lavoro minorile e il lavoro sommerso che coordino, con comunicazione del presidente Tofani, si è fatta richiesta alle prefetture delle Province della Regione Sicilia - dalla quale si è pensato di iniziare dati relativi proprio al lavoro minorile. Orbene, le stesse prefetture hanno risposto fornendo dati inutilizzabili a causa della disomogeneità dei parametri impiegati in corso di rilevazione. Questo ha reso necessaria un'ulteriore comunicazione del Presidente, allegata alla quale è stato inviato uno schema predisposto dal mio ufficio, cui le prefetture sono invitate ad attenersi.

all'incirca in linea con la percentuale dell'anno precedente. Percentuali che potrebbero da subito aumentare se, come ben rilevato dal presidente Tofani nella sua risoluzione, si riuscirà a rafforzare in maniera incisiva il coordinamento e la collaborazione fra tutti gli enti istituzionali, così come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Un dato in apparenza positivo, anche se personalmente ritengo necessiti di una maggiore riflessione, è la mancanza quasi totale del ricorso al lavoro minorile, entità numerica complessiva diminuisce nel 2009, passando da nove a tre minori impiegati, anche se tutti irregolari, a fronte di un solo minore irregolare su nove nel 2008. Ho detto in apparenza positivo in quanto il dato della prefettura di Enna è in netto contrasto con quanto lamentato da istituzioni scolastiche religiose e del volontariato in Sicilia, che ci indicano il degrado sociale in cui tutta la Regione versa a causa del continuo aumento dei tassi di dispersione scolastica, di microcriminalità e di sfruttamento del lavoro minorile. Ho inteso informarvi, peraltro solo parzialmente, sui dati pervenuti dalla prefettura di Enna a mero titolo di esempio, ma anche per sottolineare quanto sia utile il lavoro che questa Commissione e tutti i gruppi di lavoro stanno svolgendo, gruppi a cui vanno i miei ringraziamenti per quanto fatto finora. Quello della sicurezza sui luoghi di lavoro rientra nel concetto più vasto di sicurezza, da sempre tra gli obiettivi del mio partito,

la prima Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, come già sottolineato dagli altri colleghi del mio Gruppo, è frutto del lavoro unitario fin qui svolto in seno alla Commissione stessa

a sradicare nel nostro Paese quella tragedia, che in maniera a volte un po' ipocrita è chiamata delle morti bianche. Di fronte alle morti, di fronte all'invalidità, parte politica deve fare un passo indietro rispetto alle persone che vogliamo rappresentare come membri di questo Parlamento. In tal senso è doveroso da parte mia riconoscere al presidente Tofani lo sforzo costante nel ricercare posizioni condivise. Un lavoro non semplice, quello svolto dalla Commissione, che, proprio nei primi mesi della sua attività, si è dovuta confrontare con atti del Governo e della maggioranza che rischiavano di mettere in discussione conquiste condivise, frutto di anni di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. alle proposte emendative elaborate dalla maggioranza a vari provvedimenti, tese a scardinare passaggi fondamentali del Testo unico che avevano ad oggetto, ad esempio, l'eliminazione della comunicazione, entro il giorno antecedente, dell'assunzione dei lavoratori, così da mantenere in vita quella vergogna degli infortuni, anche mortali,

Un fenomeno, quello del lavoro in nero, che, oltre a riguardare ancora tanti lavoratori italiani, investe particolarmente i lavoratori extracomunitari. E, come ha giustamente sottolineato il collega Perduca nel suo intervento di questa mattina, c'è troppo poca attenzione nei confronti di questi lavoratori, che spesso operano in quei settori a maggior rischio di incidenti, anche mortali. ancora, le proposte della maggioranza tese alla cancellazione o allo svuotamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al depotenziamento dei livelli di tutela, con la deresponsabilizzazione dei naturali responsabili della sicurezza, la modifica al ribasso del sistema sanzionatorio e lo svuotamento di poteri e funzioni degli organismi di vigilanza. Non possiamo dunque sottacere una grande distanza tra i nostri convincimenti e le politiche messe in campo dalla maggioranza. Proprio in un quadro così complesso e difficile,

che avevano turbato una parte considerevole dell'opinione pubblica e che avevano interessato lo stesso Presidente della Repubblica. Devo dare atto al sottosegretario Viespoli di aver avuto la capacità di tornare indietro rispetto a testi che erano stati già presentati, mentre di solito indietro si torna raramente. Questo per dire che, di fronte ad un fatto che turbava le coscienze,

sostenuti e finanziati quegli istituti previsti dal Testo unico volti alla verifica dei controlli, sia pubblici che dei lavoratori. A tal proposito, ci preoccupa non poco un emendamento della maggioranza, approvato in Commissione lavoro, diretto a ridimensionare il ruolo e le funzioni dell'ISPEL. Il lavoro della Commissione è stato sostenuto fin qui anche da una crescente attenzione dell'opinione pubblica e dei *media* sulle quotidiane morti nei luoghi di lavoro, da tragedie che hanno scosso il nostro Paese e dai ripetuti appelli a non abbassare la guardia e a fare di più, provenienti dalle più alte cariche dello Stato, a cominciare dal Presidente della Repubblica. Le morti, gli incidenti sul lavoro, le malattie professionali non sono cataclismi naturali. E' possibile invertire la marcia, cambiare strada. È necessario anche intervenire partendo da singoli settori. Dal nostro lavoro di approfondimento e di indagine è emerso, ad esempio, che molte delle morti in agricoltura (settore ad alto rischio), ma anche in edilizia, sono dovute all'utilizzo di macchinari fatiscenti e vecchi di decine di anni. Ebbene, qui è possibile da subito assumere un'azione concreta. Il Governo si impegni, così come previsto dal dispositivo delle varie risoluzione, a prevedere misure di incentivazione alla rottamazione di macchine ed attrezzature agricole, forestali ed edili. Si faccia ora, si inserisca da subito una norma in finanziaria. Ed ancora, si traduca in norma da subito un maggiore gettito per gli enti preposti alla sicurezza e si metta freno alla rincorsa del massimo ribasso, che rischia di produrre, specialmente in edilizia, un ulteriore abbassamento dei livelli di protezione. Il Gruppo del PD, per le ragioni che ho esposto,

nelle scuole l'atteggiamento da tenere in riferimento ai luoghi del lavoro e al modo di estrinsecarlo. Che significato avrebbe sanzionare se non creiamo prima le condizioni affinché non si arrivi alla sanzione?

di produrre una serie di iniziative legislative e di atteggiamenti comuni, mettendo insieme le attività dei vari organismi che devono intervenire per la salvaguardia del posto e dell'ambiente di lavoro e per la riduzione degli incidenti sul lavoro che,

tra i vari enti istituzionali che si occupano della tutela della salute e della sicurezza del lavoro, non soltanto a livello centrale, ma anche a livello locale, determinando così un approccio univoco e coerente della pubblica amministrazione nella interpretazione delle norme e quindi nella loro applicazione. Abbiamo inoltre la necessità di mettere in essere una serie di misure di incentivazione economico-fiscale per favorire la rottamazione e la

credo che dobbiamo incentivare sempre più l'attività di prevenzione e di contrasto, in modo

e le politiche sociali*. L'integrazione riguarda un impegno nei confronti del Governo a provvedere all'emanazione del decreto del Ministro del lavoro relativo all'attivazione del fondo per i lavoratori colpiti dalle patologie correlate all'amianto. Si fa riferimento all'esigenza di monitorare e di fornire dati in relazione alla tutela dei lavoratori rispetto all'accertamento delle malattie professionali e infine ad una più forte capacità di coordinamento degli enti previdenziali per una corretta gestione del contenzioso che consenta di evitare ricorsi dilatori e concretizzi con più rapidità e certezza il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Questa è l'integrazione, sulla quale il Governo esprime parere favorevole, anche perché è stata formulata congiuntamente con i presentatori. Aggiungo anche, Presidente, proprio ai fini della votazione,

della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (*Convention on Certain relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge 7

di alcune armi convenzionali dannose o aventi effetti indiscriminati vede la più completa condivisione del Gruppo dell'Italia dei Valori. Già in numerose altre occasioni, infatti, ci siamo battuti perché l'abolizione di armi con effetti tragici come le mine, che colpiscono indiscriminatamente civili e bambini in tempo di guerra così come in tempo di pace, venisse sempre rispettata nei trattati internazionali che abbiamo siglato. Anche ultimamente lo abbiamo ricordato ai colleghi e al Governo, ossia quando abbiamo presentato un ordine del giorno sull'Atto Senato n. 1500, nel quale si stabilivano le modalità di cooperazione nel campo della difesa tra Italia ed Emirati Arabi Arabi Uniti, includendo fra le armi soggette a scambio anche le mine. Ebbene, Presidente, noi dell'Italia dei Valori, abbiamo chiesto che venissero escluse le mine dallo scambio, ma purtroppo la maggioranza ha bocciato il nostro ordine del giorno. Pertanto un Protocollo che completa l'accordo più importante in tema di armi particolarmente offensive, come quello di Ginevra, non può che vedere la nostra più completa adesione. Voglio solo soffermarmi, dunque, sul contenuto dell'ordine del giorno che abbiamo presentato alla norma in discussione oggi, recante il finanziamento del Fondo per lo sminamento umanitario. Il contenuto dell'ordine del giorno ricalca, quasi perfettamente, quello presentato dai colleghi Evangelisti e Narducci alla Camera dei deputati. I due ordini del giorno dei colleghi sono stati accolti con modifica dal Governo. In questo da me presentato ho soltanto precisato che il rifinanziamento del Fondo per lo sminamento, avvenuto finalmente con la legge n. 108 del 3 agosto scorso e riferito all'anno 2009, dalla formulazione della legge stessa pare sia limitato a sostenere economicamente operazioni di sminamento che riguardano solo i Paesi come l'Afghanistan, l'Iraq, il Libano, il Pakistan, il Sudan e la Somalia. In questo mio ordine del giorno chiedo al Governo di chiarire che l'operatività dello stesso Fondo, e quindi delle stesse operazioni di sminamento, sia estesa anche a tutte le altre aree non richiamate nella legge, cioè a tutti quegli altri Paesi che, usciti dai conflitti, si ritrovano con il territorio invaso da mine inesplose, di modo da rendere universale il prezioso supporto che possiamo dare alle popolazioni già martoriate dalla guerra, senza distinguere se sono iracheni o kosovari, così come voluto dalla *ratio* della legge 7 marzo 2001, n. 58, che ha istituito il Fondo. Chiedo inoltre, come i precedenti colleghi, il finanziamento del Fondo non sia *una tantum*, ossia per questo anno e per questo milione di euro, come si legge nella legge n. 108, e poi basta, e neppure solo per il 2010. che già ottenere il finanziamento stanziato con la legge n. 108 è stato assai difficile, chiedo che l'impegno a garantire adeguate risorse al Fondo sia per ogni esercizio annuale. Colleghi, la necessità di approvarlo - necessità umana prima che politica - è stata sottolineata con ancora maggiore rilevanza dall'ultima legge finanziaria, la quale inizialmente non aveva previsto per il 2010 il finanziamento di 1 milione di euro destinato al Fondo, finanziamento che eravamo riusciti, invece, a reperire per il 2009 nel decreto sul finanziamento missioni approvato a luglio. Essa aveva cioè, dopo soltanto 3 mesi, vanificato gli sforzi del Ministero degli affari esteri, del sottosegretario Mantica e del sottosegretario Scotti e di tutti i colleghi parlamentari in quanto, se nell'anno corrente il Fondo è adeguatamente finanziato, non lo sarebbe stato più per l'anno prossimo. Fortunatamente, grazie alla convergenza del lavoro fra maggioranza ed opposizione in 3a Commissione, siamo riusciti ad evitare, grazie all'approvazione in Commissione dell'emendamento specificamente dedicato, che la finanziaria togliesse nel 2010 quello che invece avevamo deciso di destinare per il 2009, ossia il milione di euro. Tuttavia la finanziaria non è ancora diventata legge; quindi ancora spero che non sia cosi - c'è la possibilità che le risorse trovate per il 2010 vengano cancellate. Inoltre, cari colleghi, non si può sperare che uno non si può sperare che uno strumento fondamentale per i diritti umani e per la cooperazione allo sviluppo rimanga appeso alla nostra buona volontà e alla nostra attenta vigilanza. Non ci si può accontentare del fatto che, grazie al lavoro, ottimo, della 3a Commissione, del Sottosegretario e del relatore, ogni volta si debba emendare o provvedere con un intervento normativo *ad hoc* al finanziamento del Fondo. Ecco perché vi sottolineo ancora una volta l'importanza dell'ordine del giorno, che guarda verso il futuro impegnando il Governo ad assicurare la copertura del Fondo per ogni esercizio annuale. Concordo, inoltre, pienamente con la riformulazione richiesta dal sottosegretario Scotti, recepita Scotti, recepita nell'ordine del giorno depositato in Aula. Dicono che un ordine del giorno non si nega a nessuno! Ecco, io credo che questo ordine del giorno lo dobbiamo lo dobbiamo alle popolazioni che già sono state vittime delle guerre e che ancora oggi sono minacciate dalle mine antiuomo lasciate come terribile eredità dalle guerre. Non neghiamoglielo!

Sappiamo tutti, signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, che purtroppo le popolazioni di territori interessati da guerre o da eventi bellici spesso vengono colpite duramente

Grazie,

il Protocollo V del 28 novembre 2003, relativo ai residuati bellici esplosivi.

e soprattutto ridurre i danni che possono affliggere le popolazioni dopo i conflitti. Ringrazio in questo contesto la Commissione oggi presieduta dal vice presidente Filippi, che ha dedicato molta attenzione al tema. Ringrazio anche la rappresentante del Governo, sottosegretario Craxi, ed il qui presente sottosegretario Scotti,

stata la stessa Croce rossa italiana, tramite il Comitato internazionale, a proporre di lanciare, nel quadro della Convenzione sulle armi convenzionali, un processo di negoziazione inteso a disciplinare in modo giuridicamente vincolante, e non solo con raccomandazioni, il problema dei residuati bellici esplosivi. Tali munizioni, come abbiamo detto, mettono in pericolo, feriscono e uccidono civili ancora molto tempo dopo la fine di un conflitto armato. Questi residuati bellici esplosivi rappresentano un enorme ostacolo agli sforzi di ricostruzione, oltre a colpire le persone, e rendono più difficili la fornitura dell'aiuto umanitario e la gestione o il riassetto di superfici agricole e forestali.

in Serbia e in Montenegro nel 1999, in Afghanistan nel 2001 (dove stanno purtroppo proseguendo), in Iraq nel 2003 e, infine, in Libano, dove dove sono stati fatti ulteriori appelli di peso per regolare la materia su base internazionale. Questo nuovo Protocollo, che è in vigore dal 12 novembre 2006, intende ridurre il più possibile i pericoli e gli effetti dei residuati bellici per le popolazioni civili, soprattutto mediante due strumenti. Il primo, che è il più importante per gli Stati sul cui territorio si trovano residuati bellici esplosivi, prevede l'obbligo di bonifica del territorio per quelli che hanno impiegato tali munizioni o impiegano tali munizioni esplosive, prevede l'obbligo di contribuire alla bonifica fornendo un'assistenza tecnica, finanziaria o in termini di personale. stabilisce, inoltre, l'obbligo di registrare e archiviare le informazioni riguardanti le munizioni esplosive impiegate e di scambiare informazioni allo scopo di facilitare la bonifica. Un allegato tecnico, poi, obbliga a rispettare, formulando raccomandazioni al riguardo, le direttive generali sulla fabbricazione, la manipolazione e l'immagazzinamento delle munizione esplosive.

Tra le misure sono anche previste una demarcazione delle zone a rischio e la bonifica del territorio. (che non ha una veste giuridica di vincolo, ma di raccomandazione comunque molto importante) prevede misure preventive da prendere e le procedure ottimali da applicare. alla demarcazione e alla sorveglianza come pure alla fabbricazione, alla manipolazione e all'immagazzinamento di munizioni esplosive. Concludo, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, appellandomi agli sforzi che

Signor Presidente, innanzitutto desidero aggiungere le firme della senatrice Poretti e mia all'ordine del giorno G100 del senatore Pedica, che pare non soltanto puntuale, ma anche opportuno perché rielabora alcune

investire denaro pubblico perché si possa passare allo sminamento di zone a noi vicine; penso ancora una volta ai Balcani, ma anche all'Asia centrale o al Sud-Est asiatico. Questi sono

riuscì a negoziare le fasi finali del bando mondiale delle mine antiuomo. Credo quindi sia quanto meno opportuno che l'Italia continui in questa direzione.

dedicare alla ratifica dei trattati internazionali non per recuperare il tempo passato nelle scorse legislature (che era uno degli obiettivi che ci erano stati posti in 3a Commissione permanente

sulle condizioni difficili in cui ogni volta dobbiamo presentare i disegni

È utile ricordare che l'adozione di questo Protocollo rappresenta sicuramente un evento significativo con riferimento tanto al diritto umanitario quanto al disarmo e alla non proliferazione alle armi. Più di altri, quindi,

dal collega Pedica, così com'è stato approvato in Commissione.

che riguarda la stessa materia, è incluso nella ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati nei confronti della popolazione civile. Per tali motivi, chiedo il voto favorevole dell'Assemblea.

la Commissione, la relatrice, coloro che sono intervenuti e, in modo particolare, il senatore Peterlini per l'iniziativa intrapresa. Il Governo auspica che il processo di ratifica si concluda con la massima celerità, così da consentire all'Italia - e questo è molto importante - di partecipare alla III Conferenza degli degli Stati parte del Protocollo V della Convenzione che si terrà a Ginevra il 9 e il 10 novembre prossimi. dell'*iter* riveste quindi una particolare rilevanza anche per l'immagine internazionale del nostro Paese e consentirebbe di ribadire la coerenza e la serietà dell'impegno da esso dimostrato nel settore dello sminamento umanitario. L'Italia si collocherebbe, in questo modo, nella cerchia degli Stati che danno attuazione a tutti i protocolli della Convenzione e potrebbe così partecipare a tutte le sessioni della Conferenza degli Stati parte. Come ho già detto, la ratifica va incontro a frequenti richieste della nostra società civile, cui non sfugge la forte valenza del Protocollo, sia sul piano del diritto umanitario sia su quello del disarmo e della non proliferazione. L'opinione pubblica italiana ha ripetutamente dato prova di particolare sensibilità nel riconoscere l'importanza dell'azione contro le mine e i residuati bellici esplosivi. Dopo la firma della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, risalente al dicembre scorso, la ratifica da parte del Parlamento italiano del Protocollo V conferma la linea di coerenza su cui si muove la politica estera del nostro Paese nel settore dello sminamento umanitario. Infine, voglio dare atto al senatore Pedica della piena rispondenza del suo ordine del giorno alla linea che tutti insieme, Parlamento e Governo, vogliamo seguire e quindi esprimo non un dato formale, ma una sostanziale e convinta adesione del Governo all'ordine del giorno

il mio intervento, ma ci tenevo a sottolineare che vi è una totale sintonia con quanto evidenziato dalla relatrice Marinaro e dal senatore Peterlini - che tra l'altro ringrazio

che voteremo convintamente a favore di questo provvedimento.

fatto a Roma il 3 dicembre 2008. Esso si inquadra nell'ambito della rete di accordi concernenti la navigazione marittima commerciale stipulati dall'Italia con i Paesi terzi e mira ad incentivare le relazioni tra i due Paesi, anche in vista dei progetti, in corso di elaborazione, delle «Autostrade del mare» e del «Corridoio verde». Quanto ai contenuti, la struttura dell'Accordo riproduce il modello dei Patti internazionali di specie, generalmente adottato dall'amministrazione italiana per la conclusione di accordi di navigazione con gli Stati terzi, salvo marginali modificazioni. L'ambito soggettivo di applicazione è il territorio delle parti contraenti, mentre quello oggettivo è il trasporto marittimo internazionale, con la sola esclusione delle attività legalmente riservate e, in particolar modo, dei servizi portuali e marittimi ivi specificati. Le autorità marittime nazionali competenti all'applicazione dell'Accordo sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'Italia, e l'Autorità egiziana per la sicurezza marittima. Viene sancito il principio della libertà di navigazione, onde assicurare l'effettiva applicazione dell'Accordo, oltre all'eliminazione di ogni ostacolo suscettibile di limitare l'attività delle navi di ciascuno Stato. Specifiche disposizioni sono dedicate al rispetto del principio di reciprocità nel trattamento delle navi, nonché alla disciplina degli equipaggi, delle attività marittime, di eventuali sinistri e dei redditi realizzati. Vengono altresì istituite modalità di consultazione tra i due Stati, mediante una commissione marittima mista, per assicurare l'applicazione dell'intesa, mentre il patto potrà essere modificato di comune accordo. L'entrata in vigore avverrà alla data della ricezione della seconda delle due notifiche e degli strumenti di ratifica attestante il completamento delle rispettive procedure interne e annullando e sostituendo, in tal modo, il precedente Accordo risalente al 1976. Talune previsioni sul pagamento della tassa di ancoraggio e degli altri oneri e diritti tariffari in ambito portuale sulla base del principio di reciprocità saranno effettive, su richiesta della controparte egiziana, entro un periodo non superiore a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. L'attuazione dell'Accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Quelli derivanti dalla riunione della Commissione marittima mista saranno coperti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Il disegno di legge in esame era già stato presentato nella scorsa legislatura, ma l'esame non si era concluso per

poiché l'ordinamento argentino non conosce l'istituto della condanna in contumacia, era quindi necessario disciplinare i casi di richiesta di estradizione per l'esecuzione delle sentenze pronunciate in tale fattispecie.